Nella seduta di ieri, sotto la sua Presidenza, si è verificato un caso analogo, che però ha avuto un esito completamente diverso. Ad un certo punto, lei ha messo in votazione un emendamento e, come risulta dal processo verbale, ha dichiarato che era stato approvato. Ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento, la dichiarazione di approvazione avrebbe inibito qualsiasi altra votazione.

votazione, che, una volta effettuata, ha avuto un esito completamente diverso portando alla reiezione dell'emendamento. Ciò che mi permetto di rappresentarle, Presidente, in ragione della vicinanza dei due episodi è che davvero non comprendo la ragione per la quale,

avrebbe potuto approvare se la votazione fosse avvenuta in termini di chiarezza. In conclusione, credo che sul punto debba essere fatta chiarezza, nel senso che la proclamazione del voto non può essere lasciata al buon senso di chi viene sfavorito da quel voto od al prestigio e all'autorevolezza della Presidenza. Se vi è stato un precedente ieri,

Del resto, il vice presidente Angius ha tale esperienza che è in grado di valutare sempre con molta attenzione le questioni. Faremo quindi un approfondimento, ma questo è il mio giudizio.

Signor Presidente, il Gruppo UDC utilizzerà solo cinque dei minuti ad esso assegnati per illustrare la mozione. Altri cinque minuti li impiegherò in sede di discussione.

riguarda l'eventualità che siano stati commessi reati da parte del vice ministro Visco o da parte del generale della Guardia di finanza Speciale, in riferimento all'azione da essi svolta. Questo è un accertamento che spetta al giudice penale. Vi è poi un aspetto di tipo giuridico-amministrativo, che riguarda la sostituzione del generale Speciale con altro generale a capo della Guardia di finanza. Competente a discutere di questo è il tribunale amministrativo e poi il Consiglio di Stato.

Il Senato non è organo giudiziario penale, non è organo giudiziario amministrativo, è un importante consesso politico, che ha il diritto e il dovere di discutere politicamente della questione.

da me), è stata aggiornata ad oggi perché era stata presentata a luglio di quest'anno. La ragione per la quale dopo tre mesi siamo riusciti finalmente a portare in Aula quella mozione andrebbero seriamente indagati. È la prima volta, per quello che mi risulta, che una mozione firmata dai Capigruppo dell'opposizione ha dovuto attendere un così lungo periodo. Durante l'aggiornamento dei lavori, siamo stati per così dire agevolati dal fatto che nel frattempo

deve rispondere penalmente davanti al giudice penale ed ha cominciato a farlo. Non si è conclusa quella vicenda e non mi interessa come terminerà. Il vice ministro Visco dovrà rispondere in sede amministrativa della sua vicenda. Mi chiedo perché, sino ad ora, non ha mai dovuto risponderne politicamente. Noi abbiamo una mozione, ed è la ragione per la quale i colleghi della maggioranza non possono ritenere di liberarsi della vicenda soltanto con un voto. Avrei molto piacere che ci fosse una mozione della maggioranza che mi facesse capire perché è nata questa vicenda, quando è nata, come dice l'autorità giudiziaria penale, definendo oscuri i motivi che indussero Visco a fare pressioni sul generale Speciale, allora comandante della Guardia di finanza. Quei motivi oscuri sono il fatto politico del quale dobbiamo discutere: o rendiamo chiari i motivi oscuri o non ci illudiamo che la vicenda si concluda. Nella mozione da me presentata insieme agli altri colleghi dell'opposizione si cerca di chiudere questa vicenda dando una nostra interpretazione a tale oscurità. La maggioranza, se ha un'idea diversa, la esprima, ma è importante che sappia che la vicenda, con oggi, non si conclude. Continuerà, e mi auguro che continuando anche il Presidente del Senato vorrà consentire una diretta televisiva, perché è importante che gli italiani sappiano quali sono le ragioni oscure che hanno allora indotto Visco a fare pressioni indebite sul comandante della Guardia di finanza. *(Applausi

Signor Presidente, anche in questa occasione come in quella precedente in cui già si era discusso della vicenda, anche se è intervenuto un fatto successivo alla discussione di allora del Senato, cioè

questioni che gli vengono attribuite e sulle quali il Senato oggi discute riprendendo la mozione a suo tempo presentata dal senatore D'Onofrio, illustrata poco

della procura - che, alla fine, è arrivata ad una richiesta di archiviazione a mio avviso inopinata per le motivazioni contenute nel testo descrittivo della stessa sentenza

indipendentemente, ripeto, dalle conclusioni della proposta di archiviazione che è stata posta, una valutazione di carattere politico argomentata da chi ha un ruolo al di sopra delle parti politiche,

continua, reiterata volontà di evitare di far sì che il Vice ministro renda conto e, ovviamente, paghi - com'è successo nella scorsa legislatura per altri Ministri - per le proprie azioni ed i propri comportamenti, troviamo una delle motivazioni per cui, in questi ultimi mesi e in queste ultime settimane, un grande senso di antipolitica è esploso nel Paese. Non chiediamocene, quindi, le motivazioni e non cerchiamole al di fuori di quest'Aula né solamente nel numero dei senatori o nei costi della politica; ricerchiamole, invece, negli atteggiamenti che un Vice ministro con deleghe importantissime - ha assunto e nei comportamenti che terremo oggi nel momento in cui voteremo le mozioni. Ognuno di noi ha la responsabilità della lettura dei testi: le mozioni che ha presentato la Lega sono assolutamente chiare e documentate. Ognuno di noi ha la propria

Signor Presidente, innanzi tutto vorrei osservare che la sua decisione, che ci ha comunicato ieri, di non concedere la diretta televisiva di questo dibattito mi appare francamente discutibile. E mi appare francamente discutibile la sua motivazione:

Ma di replica non trattavasi, perché le mozioni di cui discutiamo traggono, sì, origine dalla stessa vicenda (cioè l'illegittimo comportamento del Vice ministro con delega sulla Guardia di finanza), prendono spunto da un fatto nuovo, che dovrebbe essere interesse di tutto il Senato mettere in evidenza e che dovrebbe portarci a richiedere una cosa banale, ossia il rispetto della legge. Qual è il fatto nuovo? È semplice. Il giudice penale

ha definito, in modo inequivocabile e con dovizia di dettagli (come i documenti alla nostra attenzione riportano), come illegittimo.

non potrebbe essere né assegnata né congelata, ma semplicemente riassegnata al suo titolare legittimo. Invece, appare del tutto normale che il Governo, per il quieto vivere e per reggere la difficoltà dei propri rapporti,

che nella maggioranza ci hanno tormentato per anni e per tutta la campagna elettorale ergendosi, appunto, loro stessi a giudici della legalità? Signor Presidente, Presidente, ho pochi minuti e non voglio ridurmi solamente all'invettiva e alla polemica. La maggioranza ha ritenuto di non presentare alcun documento e di unirsi semplicemente nella reiezione delle mozioni presentate dall'opposizione. A me pare un segno, per così dire, forse di resipiscenza: vogliamo intenderlo in questo modo. E allora, se la maggioranza ha deciso di non mettersi in gioco con questo... un segno di furbizia, come mi suggerisce il collega Biondi, però io voglio interpretarlo come un atto di resipiscenza. E allora, siccome il Governo non si è messo in gioco in questa vicenda e non ha ritenuto di presentare un documento su cui, per così dire, chiamare la maggioranza ad un voto di sostegno, ebbene ciascuno dei senatori della maggioranza rifletta, interroghi magari la propria coscienza (se gliene è rimasta un po') e pensi che forse anche se una mozione della opposizione venisse approvata, ciò non provocherebbe la caduta del Governo, ma il ristabilirsi in quest'Aula della legittimità che manca oggi al Governo stesso.

200 miliardi di euro ogni anno; 550 milioni di euro ogni giorno dell'anno; 70 volte il costo dell'accordo sulle pensioni firmato qualche tempo fa. È questa altissima cifra che è al centro del dibattito, non altro. L'opposizione ha deciso di fare del vice ministro Visco un simbolo, tappezzando le città con manifesti dal tratto grandguignolesco, in cui egli è armato di robusti canini. Ed ora che costruiscono scientemente una occasione per sfidare quel simbolo, si accaniscono. È una strategia forse legittima, ma sfacciata, il cui vero tema del contendere sono quei 550 milioni di euro che ogni giorno vengono evasi da furbastri che ritengono che pagare le tasse sia un comportamento da sciocchi. Come già abbiamo avuto modo di discutere nella prima puntata di questo dibattito a giugno, il Consiglio dei ministri, il soggetto titolato alla nomina e alla revoca del comandante della Guardia di finanza, ha deciso l'avvicendamento del generale Roberto Speciale, essendo venuto meno il necessario rapporto di fiducia. Di fronte a criticità nell'efficacia dell'azione di taluni uffici della Guardia di finanza, la scarsa reattività del generale Speciale ha prodotto la caduta di quella fiducia che è indispensabile sussista tra autorità politica e autorità militare. Il vice ministro Visco, con grande senso di responsabilità, ha poi ritenuto di riconsegnare la delega sulla Guardia di finanza. Allora, insieme ad alti lamenti dell'opposizione, sentimmo in quest'Aula alcuni colleghi affermare che se anche Visco non si fosse dimesso, ci avrebbe pensato la magistratura. Nella metà di settembre il procuratore di Roma decide l'archiviazione delle ipotesi di abuso e minacce: archiviazione, perché il fatto non ha rilevanza penale. Noi possiamo comprendere che il giudizio politico possa esimere dalle valutazioni penali, soprattutto per una opposizione che ha nelle proprie fila diversi condannati in via definitiva per reati di una certa gravità come corruzione, falsa testimonianza e falso in bilancio. Ma conterà pur qualcosa un giudizio terzo come quello della magistratura? Le motivazioni della richiesta di archiviazione paventano possibili irregolarità amministrative. Cosa faremo allora, il Senato terrà un ennesimo dibattito se mai un giudice di pace desse ragione al generale Speciale? Questo Senato è la casa di tutti, maggioranza e opposizione, e di fronte alla richiesta perentoria dell'opposizione di un dibattito parlamentare, con senso di responsabilità la maggioranza se ne assume l'onere. Di fronte ad ogni fatto che succeda il venerdì, magari sollevato da una qualche libera testata giornalistica, puntualmente il giovedì successivo si tiene un dibattito parlamentare, con il necessario corollario di chiacchiere parapolitiche che riempiono i giornali per una settimana, e puntualmente le presunte divisioni della maggioranza si rivelano per quello che sono, pettegolezzi da *buvette*. Anche questa è una tattica tanto legittima quanto sfacciata. Non comprenderemmo le ragioni di un tale accanimento nei confronti del Vice ministro, se non ne intravedessimo le ragioni reali, cioè quei 200 miliardi cioè quei 200 miliardi di evasione all'anno che sono la palla al piede del nostro Paese, e i 10 miliardi che in un solo anno il Governo dell'Unione è riuscito a recuperare. Anche in questo caso è bene che i colleghi dell'opposizione non si facciano inutili aspettative. Se pure Visco non fosse il vice ministro con delega alle finanze - e noi ci auguriamo che egli prosegua a lungo il suo impegno - la politica fiscale della nostra maggioranza non si modificherebbe minimamente. Il centro-destra può costruire tutti i simboli che vuole, ma non riuscirà a mettere in discussione quella che è una nostra convinzione profonda: che l'evasione fiscale sia una malattia che deve essere radicalmente debellata. Confermeremo questo impegno con nuovi e maggiori investimenti per il contrasto dell'evasione anche nella prossima finanziaria. Nei primi sei mesi del 2007 sono stati scovati 300 furbastri che hanno nascosto al fisco mezzo miliardo di euro: 300 persone che devono al fisco l'equivalente della retribuzione di 20.000 lavoratori per un intero anno. Se qualcuno va a caccia dei voti di quei 300 elettori si accomodi, noi preferiamo rappresentare i lavoratori e i pensionati, che pagano le tasse fino all'ultimo euro. Come non cogliere che il richiamo alla disobbedienza fiscale, magari stemperato da rettifiche ed evocazioni di fraintendimenti, mette in discussione il tessuto sociale e civile della convivenza? Come non cogliere che, se un personaggio con responsabilità pubbliche evoca l'ipotesi di non pagare le tasse, sgretola le istituzioni democratiche? "Disobbedienza civile" è il titolo del saggio di Thoreau che ha ispirato l'azione di Gandhi e di Martin Luther King, una leva radicale per affermare il diritto all'esistenza di interi popoli. La disobbedienza civile è una forma di lotta politica, attuata da un singolo individuo o più spesso da un gruppo di pressione, che comporta la consapevole violazione di una precisa norma di legge, considerata particolarmente ingiusta; violazione che però si svolge pubblicamente in modo da rendere evidenti a tutti e immediatamente le sanzioni previste dalla legge stessa. Vedere questo estremo strumento per il riconoscimento dei diritti umani piegato alla propaganda di pagare qualche soldo in meno di tasse è un offesa a chi, in nome dei diritti umani, ha pagato in prima persona. Questo non significa, ovviamente, che il nostro regime fiscale sia ineccepibile, ma che serve serietà, rigore, responsabilità, altrimenti ci aspetta il baratro della demagogia e del populismo. Serve la responsabilità di chi, prima di abbassare le tasse, riesce concretamente ad allargare la platea dei contribuenti e a recuperare l'evasione fiscale: pagare meno, pagare tutti, e noi stiamo cominciando a dare corpo e gambe a questo *slogan*. Serve la serietà di chi sa dire anche dei no, e se le risorse non ci sono per tutte le domande, i bisogni e i desideri, è in grado di fare una scelta, a partire da chi ha sempre contribuito e, nonostante questo, non riesce, pur con il proprio dignitoso lavoro, a condurre una vita serena. Qualcuno potrà ritenere che non fosse questa la discussione all'ordine del giorno, ma purtroppo solo di questo si può discutere, vista la faziosità del tema, cioè dei motivi veri che hanno spinto l'opposizione a volere questo dibattito. Siamo fiduciosi che la maggioranza, compatta, saprà anche in questo caso dimostrare la vacuità delle presunte divisioni agitate dall'opposizione. Così come siamo certi che i cittadini sapranno giudicare e distinguere tra chi è pronto a mettere in discussione alcuni princìpi intangibili della Repubblica, come la terzietà delle Forze Armate e di Polizia, e chi, affermando il principio dell'equità fiscale, non cede alle pressioni dei soliti noti.

il vice ministro Visco era "interessato" o comunque voleva il trasferimento dei quattro ufficiali. Sul punto, non solo

e domani, qualsiasi Governo verrà in futuro, posizioni di assoluto menefreghismo circa il comportamento di un Sottosegretario, di un Vice ministro, di un Ministro che potrà essere bugiardo, fare

il nuovo dibattito sul cosiddetto caso Visco si apre in un contesto ulteriormente aggravato rispetto a quando lo affrontammo nel giugno scorso; aggravato dalle motivazioni addotte dalla procura di Roma nel richiedere l'archiviazione per l'ipotesi di reato di abuso d'ufficio e di minacce. Come è noto, e come ricordava poc'anzi il collega Franco pur riconoscendo l'inesistenza dell'ipotesi di reato, la procura ha difatti considerato illegittima la condotta del Vice ministro perché tenuta in violazione di specifiche norme che non gli conferivano il potere di disporre o di ordinare il trasferimento di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, norme di cui egli aveva consapevolezza. Infatti, prosegue la procura, «è pacifico che il vice ministro Visco abbia tentato di ottenere il trasferimento dei quattro ufficiali,

perché il potere decisionale in materia è attribuito da una norma primaria al Comandante generale. Inoltre, lo stesso documento della procura ricorda che il Vice ministro, interrogato il 24 giugno, ha parlato, a proposito dei quattro ufficiali, del loro «rapporto molto stretto con i vertici della Guardia di finanza e, presumibilmente, con la precedente «Dichiarazione - chiosano i 2 magistrati - che sicuramente confligge con i principi che nel nostro ordinamento regolano il rapporto tra autorità politica e autorità amministrativa»; Qui veniamo al punto; il rispetto dell'articolo 97 della Costituzione e dei rapporti tra potere politico e strutture burocratiche o Forze armate. Siamo convinti che il dovere del potere politico sia quello di non interferire con i compiti delle strutture amministrative, rispetto alle quali esso si deve limitare a dare direttive di carattere generale. Se si supera questo confine, si creano inevitabilmente conflitti tra organi dello Stato: questo confine, invece, il vice ministro Visco ha superato ampiamente. Non vi è nelle mie considerazioni alcun pregiudizio aprioristico; vi è solo la constatazione di una situazione che si è determinata e che ha aperto una grave frattura istituzionale. Per questo, nell'ordine del giorno che ho presentato, sottolineo la necessità, al di là di quelli che saranno gli sviluppi giudiziari e le decisioni del gip, di affidare definitivamente le responsabilità di indirizzo politico sulla Guardia di finanza al Ministro dell'economia e delle finanze. Non è più sufficiente il solo congelamento delle deleghe del Vice ministro. Occorre un provvedimento inequivocabile che serva a superare lo stato di malessere che si è determinato nei rapporti tra Governo e un Corpo essenziale dello Stato. Credo che il Governo darebbe un segnale importante, seguendo questa via, che contribuirebbe ad aumentarne la credibilità. Ma forse solamente questo non basterebbe, come indico con l'altra proposta contenuta nel mio ordine del giorno. Se vuole acquisire un'autorevolezza che oggi ha in gran parte perduto, il Presidente del Consiglio dovrebbe prendere spunto dall'episodio per procedere prontamente ad un riassetto organizzativo che conduca alla limitazione del numero dei Ministri e dei Sottosegretari, in linea con la legislazione vigente all'atto del suo insediamento, che è stata aggirata con il cosiddetto spacchettamento. Sarebbe oltretutto una risposta forte rispetto alle spinte dell'antipolitica che si stanno ormai sempre più diffondendo: una risposta che confido il Parlamento possa dare con un voto sul mio ordine del giorno che vada al di là dei tradizionali confini tra maggioranza e opposizione.

In sede di discussione, mi interessa mettere in evidenza due questioni soltanto. All'inizio della vicenda, il 16 luglio 2006

Il giorno dopo, il vice ministro Visco nella sua deposizione da indagato dice di aver parlato con il comandante generale con la bava alla bocca e di averlo preso a pesci in faccia. Vorrei soltanto capire

il ritiro della delega a Visco mi sembra perfino un fatto di buoncostume. Non lo vorrei porre in termini politici, ma è un fatto di assoluta ovvietà. Visco allora,

del vice ministro Visco sono state giudicate false dal processo penale in corso: questo è il punto politico della questione. Nel processo penale in corso si afferma che un Governo nato qualche giorno prima di questa vicenda (non anni prima) non poteva avere alcun elemento sull'evasione fiscale e che, quindi, erano del tutto inverosimili le argomentazioni usate da Visco. La parola "inverosimile" è usata nel processo penale in corso dalla procura di Roma.

Non c'entra niente la lotta all'evasione fiscale: è il tentativo sbagliato che Visco pone all'inizio della sua azione. Da allora la maggioranza continua a mostrare di ritenere intoccabile Visco per ragioni mostruosamente misteriose. Vorremmo capire le ragioni della intoccabilità fino ad ora di Visco*. Quando non sarà più intoccabile - e naturalmente ciò avverrà - è ovvio che all'interno di questa maggioranza qualcuno si chiederà perché vi è stata l'intoccabilità. È un'intoccabilità che riguarda le motivazioni per le quali Visco ha tentato di ottenere la rimozione dei dirigenti della Guardia di finanza che indagavano sul caso BNL-UNIPOL in quei giorni. Questo è il nesso politico della questione, onorevole Presidente del Senato. Non c'entra nulla la vicenda giudiziaria penale. Io sono stato costretto a modificare la mozione, aggiornandola ai dati penali, perché questi sono la prova provata della falsità delle affermazioni di Visco all'epoca, di Padoa-Schioppa quando è venuto in Aula e di questa maggioranza oggi. Prendete atto che la questione dell'evasione fiscale non c'entra nulla. Visco ha fatto quello che ha fatto per ragioni che rimangono misteriose. Vorremmo che voi chiariste una volta per tutte questo mistero. L'evasione non c'entra niente; le ragioni erano e sono politiche: riguardano l'indagine sull'UNIPOL dell'epoca e le connesse intercettazioni, argomenti sui quali quest'Aula sarà costretta a vogliate voi o no - per ragioni di ordine costituzionale. Tra qualche giorno, quando discuteremo delle intercettazioni, capiremo forse veramente qual è il nesso profondo tra la cosiddetta vicenda «Visco-Speciale» e la questione delle indagini sulla BNL-UNIPOL. Questa la questione politica che fu posta all'epoca, ad esempio, da Parisi, che riguarda il problema del rapporto tra potere politico e potere economico. Su tale questione voi dovrete fare chiarezza, caschi il mondo. *(Applausi dai

cercherò di essere breve, perché mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto sulle mozioni. Devo dire che le argomentazioni che ho sentito fin qui a sostegno di queste mozioni

perché abbiamo discusso e votato sul caso Speciale e sappiamo della rinuncia all'esercizio delle deleghe da parte del vice ministro Visco. il metodo, c'è un procedimento in corso, durante il quale è stata chiesta l'archiviazione,

Capisco che per l'opposizione esso costituisca una ghiotta occasione per «girare il fumo con la manovella», come avrebbe detto Ernesto Rossi,

Visco, nel bene e nel male, che sia simpatico o antipatico, che abbia un buon carattere o un carattere discutibile, è ormai il simbolo della lotta all'evasione ed è indicato come l'uomo nero della politica fiscale.

Noi possiamo decidere come il Presidente del Consiglio distribuisce le deleghe all'interno al Governo? È possibile impegnare il Governo a chiedere le dimissioni ad un Vice ministro? Che

resto, noi parleremo di politica fiscale. Lo abbiamo già fatto con la mozione sugli studi di settore, e senza timore reverenziale né nei confronti del Ministro né di alcune sottovalutazioni del Vice ministro.

di quei 24 milioni di lavoratori dipendenti che pagano le tasse prima di ricevere la retribuzione. Vorrei che parlassimo di questi argomenti invece di continuare a girare attorno ad una questione non

talmente chiaro che ben difficilmente la maggioranza potrà affrontarlo con lealtà in questo dibattito. Proprio in quest'Aula, oggi noi sappiamo e possiamo dire come il Governo, nella persona del Ministro dell'economia, abbia ricostruito una vicenda complessa e delicata, che metteva in gioco la credibilità delle istituzioni su uno degli affari che maggiormente hanno appassionato la stampa, l'opinione pubblica e le stesse forze politiche. Si tratta di una vicenda che ha contribuito ad innescare l'onda lunga dell'antipolitica, che lambisce le porte di questo palazzo e che poi crea i paradossi cui noi assistiamo. Ancora pochi giorni fa, il Presidente del Consiglio ci ha spiegato, in una conferenza stampa, che stiamo per ridurre i costi della politica e che probabilmente dovrà prima o poi ridurre la carica dei 103 - tanti sono gli uomini di Governo che attualmente seguono il Presidente

Amato).* Dobbiamo ragionare su quello che accadde quel giorno e su quanto accertato dalla magistratura. È molto semplice.

stato o meno bravo a gestire la leva fiscale. È stato qui difeso con delle argomentazioni e delle tesi che la magistratura ha smentito: non era vero, né presentabile l'alibi della rimozione del comandante Speciale così come ci è stato presentato dal Governo. Questo è il punto ed è per questo che le mozioni presentate hanno un'utilità,

di chiarire quali siano gli oscuri motivi - così li definiscono i magistrati - per cui casualmente il Vice ministro si sarebbe accanito proprio con quei quattro ufficiali. Provo a immaginare alcuni di tali oscuri motivi: si potrebbe trattare di una forma di avversione pregiudiziale per la Guardia di finanza quattro vittime sacrificali estratte a sorte da un cappello e quindi aggredite per un trasferimento o, più probabilmente, di un qualche legame con l'attività che svolgevano quei quattro ufficiali. Non è questo, però, oggi il punto: dovrà semmai essere stabilito da un'indagine amministrativa

anche fuori da quest'Aula e dal Parlamento, molto più delle tante questioni che sembrano appassionare i giornali. Non so se davvero il comandante della Guardia di finanza abbia compiuto atti che hanno incrinato il suo rapporto di fiducia con l'Esecutivo. Vorrei ricordare, come

che oggi dovremmo aspettarci non tanto una promessa di riduzione dei costi della politica, né un impegno generico e generalista a non ripetere trite e vecchie abitudini, abitudini, purtroppo proprie del nostro sistema politico, soprattutto quando arriva il momento di provare un impegno che in qualche modo è stato agitato, quando poi è stata l'opposizione a stracciarsi le vesti, come Caifa. Oggi dovremmo avere un Governo che dà risposte all'evidente contraddittorio che nasce tra le tesi sostenute nell'Aula e quanto in effetti è davvero accaduto. C'è poi un altro punto che non riguarda il rapporto istituzionale tra Governo e Parlamento e neppure, più in generale, il rapporto tra la credibilità dell'operato del Vice ministro e la sua permanenza in carica. La storia, infatti, non è come ce la siamo raccontata in quest'Aula: quest'Aula: è una storia che ha pesato tanto, e lo dico cercando anche di mettermi nei panni di questa maggioranza; è una storia che ha pesato proprio sulle aspettative che in qualche modo erano cresciute e si erano sviluppate e avevano portato poi, alla fine, ad un successo, seppur di misura, elettorale della coalizione che è oggi al Governo del Paese. È infatti una storia che ha squarciato dei veli e ha portato disillusioni. È una storia che ha reso impresentabile un racconto nel complesso. È un problema che giudico delicato perché nella fase che attraversiamo, che parrebbe configurarsi come una fase di transizione verso un riassetto complessivo del sistema, ciascuno deve fare un po' la sua parte, deve rassicurare quei settori della società e quei blocchi sociali che oggi non è che seguano la «serenata dell'antipolitica», ma non hanno più fiducia nella politica. È un punto che interessa tutto il Parlamento; non riguarda la maggioranza, l'Esecutivo, l'opposizione. Trascende il destino personale del vice ministro Visco che, a mio avviso, anche se si dimettesse oggi, facendo un bel gesto, non farebbe che bene a se stesso, al Paese, alla dialettica politica e, soprattutto, anticiperebbe di poco un destino che temo il Governo seguirà in blocco di qui a breve. Oggi dovremmo cercare di far capire che se si accerta incontrovertibilmente che un Ministro abusa del proprio ruolo per trasferire degli ufficiali, prima ancora che si capisca perché voleva o non voleva farlo e quanto sia o meno reato il fatto che abbia perseguito questa intenzione, amministrativamente improponibile, quel Ministro non può fare più il Ministro. Ecco il punto. È il momento di dire che un Governo nell'occhio del ciclone e che dal un punto di vista della crisi dei consensi,

il Nuovo Testamento, non so con quanta ragione storica, attribuiva ai farisei: non vuoi la promozione alla Corte dei conti? Allora ti consegno al pubblico ludibrio di un dibattito parlamentare, dove ti definisco inaffidabile. Questa roba non funziona più.

a dire che, rispetto a questa logica, il Parlamento pretende una discussione e di smascherare questo piccolo gioco dei quattro cantoni per cui l'inchiesta non era abbastanza, per cui, poiché una persona non è stata incriminata, ma è accertato che ha compiuto degli abusi dal punto di vista amministrativo, dobbiamo aspettare per vedere quanto sono gravi. nel 2001, nel 1999 o nel 1998 poteva essere una strategia. Oggi è soltanto uno spettacolo impresentabile.

Certo è che se il Ministro dell'economia, pur nella difficoltà che gli deriva dal suo ruolo di indagato davanti al Tribunale dei ministri, proprio in ragione della vicenda Speciale,

non avrebbe mantenuto il carattere di una fasulla invettiva, priva di eticità. Un'assenza di eticità, alla quale evidentemente non può portare acqua né la correttezza grammaticale, né il rinvio vuoto a princìpi di carattere generale, né tanto meno la erudita ma non colta citazione di determinate frasi, quali, ad esempio, quella di Eraclito, secondo la quale il popolo deve combattere a difesa della legge similarmente a quanto deve fare a difesa delle proprie mura. Dicevo erudita ma non colta, perché se a questa frase ne aggiungo un'altra, quella che ha chiuso il discorso del Ministro dell'economia e delle finanze, secondo la quale i fatti sono ostinati. Sotto questo profilo, probabilmente il ministro Chiti, che ha una cultura politica più vicina all'autore, potrebbe correggerle, nel senso di dire che i fatti hanno la testa dura, ma non sono ostinati. Ebbene, se dovessi fare il mio ragionamento sulla base di queste due citazioni, evidentemente la conclusione non potrebbe essere diversa da quella del definitivo congelamento delle deleghe sulla Guardia di finanza al vice ministro Visco. Di un comportamento Di un comportamento che, secondo l'intervento del Ministro dell'economia qui in Senato, era assolutamente in linea con le leggi e che invece l'autorità giudiziaria ha definito in maniera del tutto diversa. Con questo, evidentemente, non voglio dire che la politica sottostà alle valutazioni dell'autorità giudiziaria, perché questa davvero sembrerebbe una resa incondizionata, ma semplicemente che i fatti accertati in sede giudiziaria, nella loro oggettività, non possono essere privi di contenuto anche in sede politica, ferme restando alla sede politica le valutazioni conseguenti. Sotto questo piccolo profilo mi permetto di dire che nella richiesta di archiviazione, invero molto generosa, formulata dalla procura della Repubblica nei confronti del vice ministro Visco, non solo si legge che egli ha tentato di ordinare e imporre il trasferimento dei quattro ufficiali della Guardia di finanza; ciò che più importa risulta che il vice ministro Visco ha posto in essere una condotta in violazione di specifiche norme di legge, non avendo in materia alcun potere. Non solo, si aggiungeva che tutto ciò il vice ministro Visco ha fatto nella piena coscienza della antigiuridicità oggettiva dell'azione, come gli derivava da un

allora, siccome gli interventi, specialmente gli alti interventi dei Ministri in questa Aula, devono avere un senso, come riusciamo a contemperare questo accertamento di un fatto, la violazione della legge da parte del vice ministro Visco, con le dichiarazioni qui rese dal Ministro dell'economia, dell'economia, secondo le quali il buon andamento dell'amministrazione dello Stato si realizza concretamente allorquando all'unisono professionalità, assoluto rispetto delle ruoli e delle regole e inflessibile autonomia sostanzialmente sono nel senso dell'attuazione dei princìpi della Costituzione. Con un Ministro dell'economia che qui ci è venuto a dire che laddove l'assenza o anche la carenza di uno solo dei requisiti personali oggettivi che ho appena richiamato possa sostanzialmente pregiudicare la funzionalità di una branca dell'amministrazione, ne deriva evidentemente l'allontanamento di quel soggetto. Allora, questo è il primo punto in discussione, indipendentemente dagli interessi politici del momento, quasi che, ove mai si dovesse ritenere definitivo il ritiro delle deleghe al vice ministro Visco, dovesse cadere il Governo. Qui si chiede semplicemente un'operazione di coerenza, non con quello che abbiamo detto noi

Questa violazione è stata accertata dall'autorità giudiziaria, è stata conclamata in un atto che, come vedremo, tutto appare meno che ingeneroso nei confronti del vice ministro Visco. Seconda formulazione. Siamo in presenza di una persona, parlo sempre del vice ministro Visco, che, al di là dell'arroganza dei suoi comportamenti, non ha avuto esitazione nel mentire davanti all'autorità giudiziaria. Certo, da indagato ha anche il diritto di mentire, ma se questo diritto gli deriva dal suo essere indagato sicuramente è scarsamente sintonico con l'altissimo ruolo istituzionale che riveste. Perché affermo che ha mentito? Lo affermo non per mia valutazione personale ma per la valutazione che emerge esattamente da quella richiesta di archiviazione. Si legge che, in sede di interrogatorio, il vice ministro Visco, a distanza di appena un mese dal suo insediamento, avrebbe chiesto, secondo il suo dire, l'allontanamento di questi quattro ufficiali della Guardia di finanza perché poco incisivi nell'azione di contrasto all'evasione fiscale. È falso, falso, non perché lo affermo io, ripeto, ma perché l'istruttoria, gli accertamenti posti in essere dalla procura della Repubblica di Roma hanno dimostrato in maniera inequivocabile che la Guardia di finanza di Milano è stata particolarmente incisiva nella lotta all'evasione fiscale, nel contrasto al crimine economico, secondo statistiche assolutamente non comparabili con quelle di altri uffici giudiziari. Non a caso, il vice ministro Visco, scoperto in questa sua puerile menzogna, sceglie un'altra strada, per certi versi ancora più grave: quei quattro ufficiali dovevano essere allontanati perché troppo sintonici al precedente Governo, così evidentemente dimenticando la sfera di autonomia dell'amministrazione rispetto a quella della politica, ma principalmente non adducendo alcuna prova sul punto. Non solo, trovato puntuale smentita negli accertamenti effettuati dalla procura della Repubblica di Roma e principalmente proprio in quei testi, ad esempio il colonnello Ortello, che da lui stesso erano stati citati a conferma della sua menzogna difensiva.

- un signore che ha mentito spudoratamente all'autorità giudiziaria e che, soprattutto, ha posto in essere, secondo quello che dice la stessa autorità giudiziaria, un comportamento in assoluta violazione delle leggi? Potrei fermarmi

tenetevelo questo Visco, ma certo difficilmente riuscirete a spiegare tutto ciò al popolo italiano, tanto meno quelle formazioni che, al di là del nome di facciata, tutto rappresentano meno che quei valori che intendono rappresentare.

Signor Presidente, la questione che è stata posta oggi dalle mozioni e dai vari ordini del giorno è stata già affrontata e ampiamente dibattuta in quest'Aula il 6 giugno scorso, cioè il 6 giugno del corrente anno. In quella occasione il Ministro dell'economia e delle finanze illustrò ampiamente e in tutti i dettagli la ricostruzione degli avvenimenti, lasciando agli atti del Senato anche un documento scritto. Nello stesso tempo riferì al Parlamento le posizioni che, in merito a quegli stessi avvenimenti, il Governo aveva ritenuto di assumere, le decisioni prese di conseguenza. In quella occasione, in questa stessa Aula, il ministro Padoa-Schioppa spiegò anche che il vice ministro dell'economia Visco, pur ritenendo di essere nel giusto, per evitare tensioni che avrebbero potuto nuocere alle serenità degli equilibri istituzionali, aveva ritenuto di sospendere l'affidamento alla sua persona della delega sulla Guardia di finanza. Quella sospensione, com'è noto a tutti noi e a tutti voi, è operante. Da allora la delega relativa alla Guardia di finanza è tornata nelle mani del Ministro dell'economia e delle finanze e oggi niente cambia. Il 6 giugno il dibattito si concluse anche con un voto che respinse tutte le mozioni che sollecitavano interventi nei confronti del Vice ministro dell'economia, interventi che, come l'assegnazione delle deleghe, rientrano, peraltro, nella competenza del Governo. L'unico fatto nuovo intervenuto da allora ad oggi consiste nella conclusione dell'indagine condotta dalla procura di Roma la quale ha rilevato l'infondatezza dell'ipotesi di reato per la quale il Vice ministro dell'economia era stato indagato ed ha sollecitato l'archiviazione del caso; su tale richiesta dovrà ora pronunciarsi il GIP. Francamente desta perplessità che sia stato sollecitato un nuovo dibattito dopo la discussione e il voto di giugno scorso e dopo la chiusura dell'indagine della procura con la conseguente richiesta di archiviazione per l'insussistenza dei reati ipotizzati. Le mozioni presentate fanno in particolare riferimento ad alcune affermazioni contenute nelle richieste di archiviazione presentata dalla procura della Repubblica di Roma. Ma commentare in questa sede quelle affermazioni, trarne giudizi o contestarne i significati e le implicazioni non credo che sia opportuno per il rispetto stesso verso la funzione giurisdizionale. Tra l'altro siamo in una fase processuale non ancora conclusa in quanto la richiesta di archiviazione è un semplice passaggio di una procedura giudiziaria in corso. È quindi sbagliato formulare giudizi fondati su valutazioni che non hanno ricevuto nessun riscontro, oppure si vogliono far derivare conseguenze istituzionali concernenti l'assetto dei Governi da un provvedimento giudiziario assolutamente provvisorio che, peraltro, almeno nel suo dispositivo, esclude ogni responsabilità? È tutto questo conforme ad una minima esigenza di garantismo che non può essere richiamata a giorni alterni a seconda di chi riguarda o risponde forse alla necessità di autonomia e di responsabilità da parte della politica? Ma oggi, in quest'Aula del Senato, in realtà, se a questo confronto si vuole dare un senso che superi la pura e semplice strumentalità, io credo si stia tentando anche di mettere in discussione nei fatti, oggettivamente, attraverso la figura del vice ministro Visco, anche un altro tema, peraltro evocato in alcuni passaggi delle mozioni dell'opposizione, anche se non ora nel dibattito, e cioè la politica fiscale del Governo che, giustamente, alcuni esponenti della maggioranza hanno richiamato. In questo contesto allora non posso non ricordare il ruolo fondamentale che il Vice ministro dell'economia ha svolto nell'ambito dell'azione di recupero di gettito fiscale evaso portata avanti dal Governo, con risultati che non hanno precedenti. Sia pure tra mille difficoltà e ostacoli quel lavoro sta superando, mese dopo mese, ogni previsione. Esso ha fornito un contributo decisivo perché i conti pubblici del Paese potessero registrare un miglioramento più rapido di quanto i vincoli comunitari ci richiedevano e perché, proprio con la legge finanziaria appena presentata al Parlamento, che stamani il ministro Padoa-Schioppa ha qui illustrato, sia stato oggi possibile intervenire concretamente con un sostegno economico a favore dei più deboli, avviare una riduzione dell'onere fiscale sulle famiglie, ridurre l'ICI, aiutare gli italiani che pagano un affitto e approvare le riforme che introdurranno, insieme ad un notevole taglio delle aliquote IRES e IRAP, una straordinaria semplificazione fiscale per le grandi e le piccole imprese. In particolare, nel 2006 il gettito erariale è cresciuto, rispetto all'anno precedente, di 35,8 miliardi di euro; di questi, 10,8 sono frutto della crescita dell'economia, 8,1 derivano dalle vecchie *una tantum* e 5 sono il risultato di manovre permanenti. Il resto (cioè circa 12 miliardi) deve essere imputato alla lotta all'evasione: il decreto emanato nel luglio 2006 ha permesso un recupero di 2,4 miliardi e ve ne sono altri 9,5 che, sempre nel 2006, non trovano altra spiegazione se non nell'emersione spontanea di redditi che in passato erano stati occultati a fini tributari. Per il 2007, la finanziaria prevedeva norme contro l'evasione e l'elusione fiscale, sulla base delle quali si è stimato un incasso strutturale di altri circa 7 miliardi di euro. Anche quest'anno si sta registrando una quota di gettito che va ben oltre queste previsioni e che supera di gran lunga il normale aumento delle entrate dovuto alla crescita economica. I progressi compiuti nel recupero strutturale di gettito dall'evasione fiscale sono dunque imponenti, tali da cominciare ad intaccare in modo serio un fenomeno da tutti considerato pandemico. Si tratta di cifre che non lasciano spazio a dubbi sull'efficacia dell'azione svolta da questo Governo sul fronte fiscale, anche grazie al lavoro del Vice ministro in carica e di tutti i soggetti impegnati, compreso, ovviamente, l'impegno forte, attento e positivo della Guardia di finanza. Ma il recupero dell'evasione è solo un aspetto. È importante ricordare anche ciò che, attraverso la legge finanziaria appena presentata, si sta facendo per la semplificazione degli adempimenti previsti per le imprese: un milione di piccoli imprenditori potrà liberarsi dei libri contabili, della partita IVA; senza l'IRAP, avrà un solo adempimento a *forfait*. E questo avrà ripercussioni anche sull'avvio di piccole imprese da parte dei nostri giovani, con minori ostacoli. In conclusione, su questo specifico aspetto della politica fiscale, nelle condizioni in cui oggi si trova il Paese, l'efficacia e la competenza nella gestione di questa materia sono risorse importanti, e tali dovrebbero essere considerate da chiunque abbia a cuore non soltanto il buon andamento dei conti pubblici, ma anche il risanamento della piaga economica e morale dell'evasione fiscale. Questa battaglia ha come meta la riconquista di un corretto funzionamento dei mercati, grazie al contrasto fermo e deciso della concorrenza sleale praticata da chi non paga il dovuto, facendone ricadere gli oneri su chi si comporta in maniera onesta e corretta. Da ciò dipende il consolidamento di condizioni essenziali per l'espansione dello sviluppo e per la crescita economica del Paese, ma anche per il recupero della credibilità delle istituzioni e della fiducia in esse da parte dei cittadini. Si parla tanto e giustamente di legalità in questo periodo: la legalità economica ne è un aspetto fondamentale. Per questi motivi (questo secondo, legato alla politica fiscale del Governo e al ruolo del vice ministro Visco, e il primo, legato a cosa non vi è di nuovo, e cioè niente rispetto al 6 giugno), esprimo il parere contrario del Governo rispetto alle mozioni e agli ordini del giorno in discussione. Ritengo così di aver illustrato i motivi di questo parere contrario.

Presidente, colleghi, le mozioni presentate oggi dall'opposizione mirano a revocare definitivamente le competenze del vice ministro Visco sulla Guardia di finanza e a chiedere nel contempo le dimissioni di questi da Vice ministro dell'economia e delle finanze. Per poter affrontare con la dovuta attenzione l'argomento, è importante ricordare che ci troviamo a svolgere questo dibattito solo perché, immediatamente a margine della richiesta di archiviazione del caso Visco della procura di Roma, talune voci della maggioranza, per altro isolate, hanno voluto riaccendere il fuoco su vicende passate e già dibattute in quest'Aula. Nella logica dell'opportunità politica, infatti, è da giudicare inappropriato, secondo quelle voci, non sottoporre a valutazione chi ha violato la legge. Ma il punto focale è proprio nel voler ricercare a tutti i costi una violazione di legge che non c'è stata, offrendo in tal modo all'opposizione una ghiotta occasione per avanzare mozioni di sfiducia individuale

dovendo preoccuparsi di fronteggiare mozioni-stangate, la cui unica ragione risiede nel far leva sull'attuale risicata maggioranza di questo Senato. L'ho sostenuto mesi or sono e lo ribadisco adesso: la lotta e le polemiche pretestuose dell'opposizione contro questo o quel parlamentare, questo o quel provvedimento hanno l'unico scopo di montare una contrapposizione tra istituzioni dello Stato, avvelenando avvelenando il clima politico del nostro Paese. Il dibattito odierno non è altro che l'ennesimo espediente provocato dal centro-destra, con l'aiutino di turno di qualcuno all'interno della maggioranza, che è riuscito a calendarizzare le suddette mozioni sull'operato di Visco. Davanti a tali pretestuose manovre di una opposizione che ambisce solo allo sfascio istituzionale, siamo chiamati ancora una volta a dare un nuovo rinforzato segnale di coesione e fermezza. Per questo oggi i Popolari-Udeur voteranno no alle mozioni nn. 124 e 141. Signor Presidente, colleghi, il senatore Storace appena lesse che forse sarebbe stato indagato si dimise subito da Ministro della salute per sapere, 7 mesi dopo, che niente era a suo carico. Il vice ministro Visco ha emanato un atto illegittimo, violando chiaramente il precetto (come dice la procura della Repubblica di Roma) e non ha pensato minimamente a dimettersi, e questo credo che si commenti da solo, perché la statura politica e morale delle persone e degli esponenti politici si vede proprio da questi atti e da questi comportamenti. Il popolo italiano è stanco, molto stanco di questi comportamenti, perché davanti alle malefatte incredibili e inammissibili che questo Governo e i suoi singoli esponenti commettono, l'italiano, il cittadino medio è chiamato, un po' come diceva Totò, a pagare sempre e solo. Ma è ora che paghiate un po' voi, signori del Governo, e in questo caso paghi lei, signor Vice ministro, che non ha neanche il decoro, il buon gusto, il coraggio, la dirittura morale di presentarsi in quest'Aula e assumersi le proprie responsabilità davanti all'Assemblea del Senato. I suoi comportamenti sono illegittimi, ma per per le sue contraddizioni, i suoi provvedimenti vessatori, i suoi insuccessi, la sua impopolarità, la sua arroganza e la sua alterigia è ora che, anche per questi motivi, ella si faccia da parte. parte. Certo, questo è un dibattito che si concentra sulla vergognosa rimozione del generale Speciale, un integerrimo servitore dello Stato a cui va tutta la solidarietà e la stima della destra italiana. Ma purtroppo questa è solo la punta dell'*iceberg*, perché la vostra politica economica fatta di tesoretti occultati, di spesa pubblica fuori controllo, di tassazione selvaggia, di emergenza finanziaria che per la prima volta ha visto addirittura aumentare il prezzo del pane è ormai vergognosa e insopportabile. Un Governo pieno di contraddizioni, diviso su tutti, pieno di veti incrociati su tutto, ma che in questo caso stranamente si appresta ad essere più che mai "unito" o meglio UNIPOL, perché solo faccende losche ed intrallazzi vi compattano, cari amici della maggioranza. Allora, rivolgendomi ai tanto onesti colleghi, agli integerrimi magistrati: chiarite una volta per tutte da che parte state, perché questa volta è in discussione sul banco la moralità dei comportamenti di ognuno di noi. Oggi certo, è in discussione la revoca definitiva delle deleghe del vice ministro Visco e non vogliamo, per comportamento, per correttezza, per rispetto di quest'Aula dirle quello che vorrebbe dirle

troppe illusioni, perché la revoca delle sue deleghe e di quelle di tutto il Governo Prodi arriverà tra poco e definitivamente da parte del popolo italiano.

un modo di procedere invalso nel Senato, quando lei ha ricevuto l'applauso dopo il suo intervento, io ho applaudito per parti separate, nel senso che ho applaudito il passaggio in cui faceva riferimento all'oggi niente cambia - poi ci ritornerò avrei applaudito con minore enfasi quello che è venuto dopo. Mi preme in quest'Aula fare un ragionamento con la nostra maggioranza, in cui è l'Italia dei valori, e con il nostro Governo, in cui è l'Italia dei valori, non avere prima rimarcato che arriviamo a questo dibattito non perché - come qualcuno ha detto prima di me ci sia stata volontà da parte di alcune frange della maggioranza: è tutta la maggioranza che ha favorito il dibattito, forse incalzata da qualche forza più sensibile, ma se ci fossimo arroccati, probabilmente i senatori Palma o D'Onofrio non avrebbero potuto dire le cose che hanno detto in quest'Aula. Proprio perché pensiamo che questa maggioranza non si debba mai arroccare, abbiamo favorito nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi qui in Senato che si arrivasse al dibattito, non perché fosse inutile - non lo riteniamo inutile perché oggi il Governo ha detto qualcosa - ma anche e soprattutto perché la maggioranza che interessa all'Italia dei valori è una maggioranza che non si arrocca.

la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato e resteremo in questa maggioranza fino a quando queste condizioni esisteranno. Perciò - dicevo - ho applaudito per parti separate. Sta di fatto che si discute perché noi della maggioranza abbiamo voluto che si discutesse e sta di fatto che il rappresentante del Governo, di cui fa parte l'Italia dei Valori, oggi afferma che quello che l'Italia dei valori aveva richiesto in tempi non sospetti, quindi prima della polemica della polemica pubblica, prima di tutto quanto poi è avvenuto e avverrà ancora nelle aule giudiziarie, sembrava essere un fatto di evidente logicità: il rapporto incrinato tra cittadini ed istituzioni, perché c'era un comportamento non comprensibile. Rispetto a quel comportamento non comprensibile avevamo sollecitato che si ponesse fine ad una situazione di difficile comprensione da parte dall'elettorato, questo è avvenuto,

elettori, popolo e Governo; pensavamo che il Governo dovesse dire esattamente quello che ha detto il ministro Chiti, cioè che oggi nulla cambia rispetto alle deleghe che sono ritornate in capo al

perché è un Governo in cui si dimostra ancora che si ha a cuore l'interesse pubblico più che quello privato ed è un Governo che prende atto del fatto che quelle deleghe in capo al ministro Padoa-Schioppa debbono restare in capo al Ministro delle finanze, così come peraltro in quarantacinque anni di vita repubblicana è sempre avvenuto. Pensiamo che le cose dette qui dal ministro Chiti siano le condizioni che ci consentono di respingere come strumentali

...abbiamo consentito il dibattito. Abbiamo consentito che in Aula si potessero dire le cose che ciascuno di noi ha detto, nella consapevolezza che solo quando i problemi sono affrontati apertamente probabilmente si riesce a trasmettere fiducia a coloro in nome dei quali abbiamo chiesto ed ottenuto voti e fiducia e rispetto ai quali non si potrà mai dover usare come argomento di spiegazione «lo hanno già fatto gli altri prima». Siamo qui per fare cose diverse da quelle che hanno fatto gli altri prima.

intanto con una descrizione dei fatti. Abbiamo sentito la necessità di essere qui, nuovamente, per riaffrontare la vicenda Visco-Speciale, poiché non condividiamo gli esiti che ne sono derivati, non certamente rispetto al giudizio della magistratura. Riteniamo che proprio il giudizio di quest'ultima non possa non consentire altro che l'allontanamento da quelle responsabilità del vice ministro Visco. Siamo, infatti, ancora fermi sulle nostre convinzioni e insieme a noi anche molti italiani, come risulterà al ministro un certo comico, dai dati di alcuni sondaggi fatti dai maggiori quotidiani italiani. Da questi sondaggi emerge chiaramente che gli italiani ritengono che Visco avrebbe dovuto dimettersi, che la cacciata di Speciale sia stata un errore e che l'intera vicenda sia stata gestita in maniera assolutamente poco trasparente da questo Governo. Insomma, è inutile nascondere che l'intera compagine governativa non sia uscita affatto bene da questa incresciosa vicenda. Ricordiamo il sorriso del ministro Padoa-Schioppa e gli insulti che frammistava al generale Speciale, che risulta parte lesa anche dal giudizio della magistratura. La richiesta di archiviazione non soddisfa né convince, anche perché le scelte politiche, dietro le quali Visco si è trincerato a giustificazione del suo gesto, vivono di "opportunità" e ponderazione, doti del tutto assenti in tutta questa vicenda. Se Visco non è in grado di valutare opportunamente le sue decisioni, le sue scelte, è suo dovere dimettersi e il fatto che ciò non sia avvenuto avvalora ancor di più la nostra tesi. Visco non è in grado di capire cosa sia opportuno e saggio fare per l'intera immagine del suo Governo? E allora sia il Governo stesso ad agire, a tentare di recuperare un po' di fiducia nell'opinione pubblica. Ma anche questo sarebbe saggio ed opportuno, e invece siamo noi dell'opposizione, nel tentativo di salvaguardare le istituzioni del nostro Paese, a dover chiedere nuovamente un atto quasi dovuto. Non credo che in altri Paesi ciò sarebbe stato necessario. Fortunatamente, anche all'interno di questa maggioranza vi è chi condivide le nostre preoccupazioni, ma la sua voce viene stranamente tacitata, soffocata dai molteplici interessi coinvolti. Tace pensando di salvare la faccia a questo Governo, senza rendersi conto che ormai vi è poco da salvare. La vicenda di certo ha posto lo spunto per una seria riflessione, sia sui non sempre agevoli e limpidi rapporti tra il potere politico e quello militare nel nostro Paese, sia sullo *spoils system*, che la stessa Corte costituzionale, con le sentenze nn. 103 e 104 del 2007, ha definito sostanzialmente contrario alla Costituzione. L'*escamotage* proposto dall'Italia dei Valori al Governo, per superare lo scoglio di questa vicenda, non ci convince: proporre il congelamento delle deleghe a Visco equivale a condannarne il comportamento. Allora, perché esitare fino a dopo la finanziaria e l'approvazione della legge elettorale? Se Visco ha sbagliato - e noi diciamo che ha sbagliato - allora gli si revochino le deleghe e rassegni le proprie dimissioni; e si cerchi di agire in modo coerente con i propri convincimenti. È infatti questo quello che chiediamo oggi qui: coerenza, chiarezza, responsabilità, ripristino della dignità delle nostre istituzioni, sia politiche che militari. Non e' possibile, ministro Di Pietro, ammettere ma tentare di conservare lo *status quo*. Le vicende politiche dei nostri giorni non ammettono *impasse* di alcun genere; ad essere in gioco ci sono valori e interessi troppo alti, che prescindono dalle vicende dei singoli. La questione non è più solo politica e questa è oramai opinione comune. Il cittadino non crede più nelle istituzioni e nella buona fede della propria classe dirigenziale e politica. Credo che sia una grave sconfitta per tutti noi che qui, in quest'Aula, li rappresentiamo. Se viene meno anche la fiducia nelle Forze dell'ordine, poveri noi, poveri cittadini. La vicenda giudiziaria si è archiviata per un cavillo, ma non altrettanto possiamo fare noi a livello politico. Per noi che ogni giorno affolliamo quest'Aula, rilevano più i comportamenti illegittimi, anche se non penalmente rilevanti. Siamo politici e parlamentari, non giudici; non assolviamo Visco, ma lo condanniamo, Come la stampa ha giustamente denunciato, «illegittima, illecita o indebita, le sfumature delle parole non cambiano la sostanza e cioè che la condotta tenuta dal vice ministro Visco non è tollerabile per chi rappresenta le istituzioni». Infatti per noi non è tollerabile.

oggi voteranno per le non dimissioni del vice ministro Visco. Come mai? Bisogna che questi italiani si sveglino e guardino a chi si rivolge a loro

Il silenzio del Governo e della sua maggioranza ci inquieta e ci imbarazza come italiani, ci delude come cittadini. Come poter difendere la funzione svolta dalla politica dagli attacchi continui di cui siamo vittima davanti a situazioni come queste? Avrebbero ragione i nostri detrattori solamente se anche noi rimanessimo in silenzio, avallando comportamenti illegittimi in un mutuo scambio di compiacenze. Il dispotismo non può essere tollerato, né rinchiuso in un fascicolo giudiziario. Per questi motivi, per il desiderio di riportare il cittadino vicino alla politica, per riconquistare la sua fiducia verso le istituzioni,

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con le dichiarazioni in quest'Aula del ministro Vannino Chiti noi riteniamo che la questione sul caso Visco sia superata. Forse sarebbe valsa la pena che il Senato non tornasse ad impegnare un'intera seduta pomeridiana a discutere di un caso del quale avevamo già dibattuto a metà di giugno. Di certo sarebbe stato più proficuo impegnare questo tempo per parlare della politica finanziaria ed economica, della quale dovremo occuparci nella prossima legge finanziaria. e visto che siamo stati nuovamente chiamati ad affrontare questo argomento, noi crediamo che le dichiarazioni del ministro Chiti sul fatto che le deleghe per la Guardia di finanza restano nelle mani del ministro Padoa-Schioppa rappresentino la soluzione che contribuisce a rasserenare gli animi e ad evitare ulteriori strumentalizzazioni da parte dell'opposizione. Come Gruppo Per le Autonomie siamo soddisfatti che il Governo abbia recepito questa che era una delle nostre proposte, già formulata nel dibattito sul caso Visco-Speciale, svoltosi in quest'Aula a metà giugno. In quell'occasione, signor Ministro, avevamo ribadito anche l'importanza che la procura della Repubblica potesse svolgere il proprio lavoro in piena serenità. Di fatto la procura di Roma ha chiesto l'archiviazione delle ipotesi di reato di abuso d'ufficio e di minacce per il vice ministro Visco, in quanto la sua condotta è stata ritenuta illegittima ma non illecita, con una formula - diciamo così difficile da comprendere anche a chi è giuridicamente attento. Tuttavia, il giudice per le indagini preliminari non si è ancora pronunciato sulla proposta di archiviazione fatta dalla procura di Roma. una maggiore conferma dell'inopportunità di questo dibattito, che si inserisce praticamente in un *iter* giudiziario ancora non concluso.

In tal senso, indichiamo sistemi europei come quelli dell'Austria, della Germania e della Svizzera, dove l'obiettivo è quello di creare una cultura contributiva corretta, finalizzata ad un fisco non persecutorio ma sempre più amichevole. Ricordo per inciso che già la parola

le piccole e le grandi, accompagnandole e concordando con loro momenti di consultazione preventivi alle stesse sanzioni; solamente quando poi, nonostante le consultazioni e gli avvertimenti, le aziende proseguano nelle irregolarità, scattino le sanzioni.

richiesta di mantenere le deleghe in capo al Ministro stesso ci fa ritenere superflue e strumentali le mozioni proposte dall'opposizione. Pur contenendo alcune delle nostre stesse proposte, riteniamo che tutte queste abbiano come unico e solo obiettivo quello di mettere in crisi il Governo. Per questo motivo, rassicurato dalle parole del ministro Chiti, a nome del Gruppo Per le Autonomie preannuncio il nostro voto contrario alle mozioni e agli ordini del giorno dell'opposizione. Colleghi,

Mi pare però sia già in atto una modifica, nei fatti, del sistema bicamerale. In questo ramo del Parlamento si svolgono discussioni politiche, discussioni di politica generale che si concludono con mozioni e ordini del giorno: solo in questo ramo del Parlamento. L'opposizione è ancora alla ricerca della spallata, che finora non si è realizzata. Certo, con questi numeri l'incidente

davvero pensa l'opposizione di mettere in crisi il Governo con un ordine del giorno oppure con un ordine del giorno tranello del senatore Calderoli?

nei confronti del vice ministro Visco, che è il massimo artefice, ritengo, della lotta all'evasione fiscale e uno dei pilastri della finanziaria che discuteremo nei prossimi giorni. È surreale che, a fronte di una richiesta di archiviazione, l'opposizione si comporti come se sussistesse invece una richiesta di rinvio a giudizio. Noi riconfermiamo la nostra fiducia e stima nei confronti del vice ministro Visco nei confronti della Guardia di finanza, per il ruolo importante che questa svolge contro l'evasione fiscale, per la prevenzione e gli accertamenti fiscali, per il controllo delle frontiere contro il contrabbando, per la prevenzione e gli interventi relativi all'immigrazione clandestina. Quella relativa alla sostituzione del generale Speciale è stata una vicenda

e veleni. Con i sospetti e i veleni non si rende un buon servizio alla democrazia, alla trasparenza, al rigore, alla correttezza dei comportamenti, alla separazione e all'autonomia dei poteri dello Stato.

stanco e si allontana dalle istituzioni e dalla politica. Una pronuncia della magistratura stabilisce che il vice ministro Visco non ha compiuto atti penalmente rilevanti, ma atti che potrebbero essere rilevanti sul piano civile. Ma noi ci chiediamo: quali atti ha compiuto il vice ministro Visco? Visco? Telefonate? Conversazioni? Sollecitazioni? Arrabbiature? Quali atti? Noi ribadiamo la nostra fiducia nella magistratura penale, civile, contabile, ma ci chiediamo quali atti siano stati compiuti. Il Vice ministro è forse antipatico a qualcuno? Lo si dica. È troppo rigido nella lotta all'evasione fiscale? Lo si dica. Su questo punto si potrebbe certamente discutere (e lo abbiamo già fatto), non sulle ricostruzioni complottistiche e poco trasparenti, delle quali non siamo disposti a discutere. Ora l'opposizione chiede di rendere permanente la revoca al vice ministro Visco delle competenze relative alla Guardia di finanza. Abbiamo ascoltato in questi anni grandi lezioni di garantismo, molto spesso un po' pelose. Infatti ci chiediamo: perché rendere permanenti le revoche, quando la magistratura non si è ancora espressa definitivamente? Non condividiamo Non condividiamo queste posizioni ma ci rimettiamo al parere del Governo, sperando che questo, nella sua autonomia e responsabilità, e come avvenuto precedentemente, respinga decisamente questa proposta.

i fatti contestati a Visco non riguardano misure di lotta all'evasione fiscale? O invece al contrario, i trasferimenti di alcuni ufficiali della Guardia di finanza riguardano proprio

solo per la credibilità del Governo, ma anche perché verrebbe messa in discussione la linea della lotta all'evasione fiscale: per questo noi chiediamo di respingere le mozioni Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, questo inutile dibattito è stato voluto da una maggioranza che si è formata nella Conferenza dei Capigruppo fra i Gruppi del centro-destra e l'Italia dei Valori. Tempo sprecato del Parlamento, occasione di propaganda per l'opposizione: pazienza. Ora l'Italia dei Valori alla furia francese ha fatto seguire la ritirata spagnola: forse dovranno occuparsi di altri eventi rilevanti accaduti in giornata, per esempio l'arresto del capogruppo dell'Italia dei valori alla Provincia di Genova, con l'accusa di peculato e accesso abusivo al sistema informatico aggravato in quanto pubblico ufficiale. In ogni caso, avendo apprezzato le dichiarazioni del ministro Chiti, il Gruppo della Sinistra Democratica voterà contro tutte le mozioni che sono state presentate.

che il Vice ministro ha illegittimamente effettuato pressioni sul comando della Guardia di finanza per gli avvicendamenti a Milano? CORO DAL che ha mentito alla procura della Repubblica, cercando di negare tali vicende e cercando di giustificare questo proprio intervento con delle motivazioni dichiarate, Allora, signori, se queste cose sono vere (cose sulle quali il ministro Chiti ha glissato in maniera poco opportuna e sulle quali anche altri colleghi, come il senatore Formisano, hanno cercato di non dare risposta), la veridicità di queste due affermazioni induce indubbiamente ad un giudizio politico molto grave che, a mio avviso e ad avviso della Lega Nord, e secondo le mozioni presentate, dovrebbe condurre alle dimissioni o, perlomeno, all'allontanamento di questo Ministro. *(Applausi dal

grazie e complimenti, anche perché avete detto che chi conduce la lotta all'evasione, chi riscuote tanti soldi dai cittadini, alla fine può anche forse transigere a determinate condizioni di correttezza amministrativa e funzionale. una rapina a mano armata del vice ministro Visco nelle nostre tasche, nelle tasche degli imprenditori, a vostro avviso è legittima: in effetti è quanto accade. Bravi e complimenti! La procura della Repubblica ha scritto tantissime cose che dimostrano questo: avete fatto finta di non leggerle, vi affidate solo a delle conclusioni, ma esiste comunque

le conosciamo: le motivazioni si chiamano UNIPOL, si chiamano interessi nel controllare magari certi tipi di evasioni più o meno occulte, evasioni fiscali di cui il Vice ministro si erge a paladino. Vorrei anche chiedere al Vice ministro, se si degnasse di essere presente, di dirmi qualcosa sull'evasione multimiliardaria da parte delle concessionarie dei monopoli di Stato o magari se erano di suo interesse le domande fatte nell'ambito delle indagini sulle *slot machine*. Quale galassia ruota attorno a questi enormi *business*? Qui, signori, vi è la risposta dell'interessamento del vice ministro Visco, risposta che la procura non ha saputo dare nei confronti dello spostamento degli ufficiali della Guardia di finanza di Milano. Allora, non solo possiamo constatare che le conclusioni dell'indagine danno del bugiardo a questo Vice ministro (leggete e lo vedrete in maniera chiara ed inequivocabile), ma credo che, di fronte ad una di fronte ad una evidenza di questo tipo, per motivazioni proprio comportamentali, siamo obbligati seriamente a chiederne le dimissioni. L'antipolitica si nutre di queste insufficienze, di questa impenitenza di chi si permette di mentire spudoratamente, nascondendo i veri obiettivi delle delle proprie azioni. Però, alla fine, Visco salva se stesso; voi salverete Visco e con questo sarete pari responsabili di quanto ha fatto. Lo giustificate. Quindi, sia ben chiaro che dovete vergognarvi come dovrebbe fare lui.

affermando correttamente che il suo comportamento aveva minato il rapporto di fiducia che deve sussistere tra lo stesso Vice ministro e il Corpo della Guardia di finanza. Che fine fanno oggi queste affermazioni? Cos'è? È stata erta una trincea di fronte alla semplice garanzia che non verranno restituite le deleghe sulla Guardia di finanza? È compatibile la posizione che abbiamo sentito da parte del collega Formisano, con le affermazioni di poco tempo fa del ministro Di Pietro, con la politica delle mani pulite, con la quale vi riempite la bocca a giorni alterni nei confronti di chissà cosa e chissà chi e non certo del vostro Governo?

poco più di battute o dei luoghi comuni, ha avuto il consiglio e il modo, l'accortezza sua personale - cui va dato merito - di dimettersi da Sottosegretario. Ma è evidente che a voi queste cose non importano e il vostro comportamento sta dimostrando un atteggiamento

oggi individuiamo una delle tante motivazioni, ma che questo fenomeno sia coniugato ad un insufficiente livello culturale dei cittadini è un'affermazione ridicola e ignorante, offensiva della dignità dei cittadini stessi, senza riscontro alcuno, se non nella mente malata di chi ha pronunciato quelle frasi. *(Applausi dal Gruppo

molto contenute). Se il Ministro avesse rivolto a qualsiasi altra Regione le stolte e deliranti frasi che ha pronunciato nel Veneto, se avesse offeso tutti i siciliani a causa della mafia o gli altoatesini per la cultura tedesca, per quanto riguarda

per piegare a proprio uso e consumo la Guardia di finanza e offende i cittadini con opinioni gratuite e insussistenti. Colleghi senatori, anche a fronte di queste ultime osservazioni vedete se volete assumervi la responsabilità di mantenerlo al suo posto.

in questo momento al Senato si compone di almeno tre parti: il rapporto tra maggioranza e opposizione; questioni interne alla maggioranza di Governo, come risultato dagli interventi dei colleghi Barbato e Formisano poco fa; la questione specifica del rapporto tra Visco e Speciale. Parto da quest'ultima, perché vorrei dire, mi auguro per l'ultima volta, che al Gruppo UDC non interessa per nulla la vicenda giudiziaria del rapporto Visco-Speciale. Vorrei fosse chiaro che noi, fin dal primo momento, abbiamo cercato di impostare una questione politica che fino ad ora non ha avuto alcuna risposta.

del cosiddetto caso Visco-Speciale e quindi il dibattito, con oggi, comincia ad affrontare il problema. Lo dico perché i colleghi della maggioranza che sono intervenuti sappiano saranno indotti o costretti ad ascoltare ancora una volta tale questione, che non ha nulla a che fare con i problemi giudiziari di Visco e di Speciale ma con il problema politico dell'indagine giudiziaria e fiscale sull'UNIPOL, di che cosa questa rappresentava all'epoca, perché all'epoca è stata considerata un fatto di rilievo politico notevole e perché è scomparsa improvvisamente, ammantata, per così dire, di vicenda giudiziaria.

Se dovessimo fare gli interessi dell'opposizione dovremmo dire: «Tenetevelo a lungo: più a lungo Visco sta al Governo meglio le cose vanno per noi dal punto di vista elettorale». Ma non è questo il problema. non è questo il problema. Abbiamo già condotto questa battaglia politica nei confronti di Visco e la questione la considero da tale punto di vista ripetitiva. Il problema era e rimane

illegittimità di un comportamento conseguente ad un fatto specifico, cioè l'interferenza illegittima nei poteri della Guardia di finanza. Non è un fatto di poco peso, colleghi della maggioranza, è una questione dirimente: se un Governo ha al proprio interno

della natura del rapporto tra potere di governo e potere economico del nostro Paese. Non è questione banale; c'è stata nella prima Repubblica e nella cosiddetta seconda Repubblica e rileva anche dal punto di vista politico dei rapporti tra il nascituro Partito Democratico e il potere economico del nostro Paese.

Colleghi, io vorrei concludere le dichiarazioni di voto,

mi porta alla memoria una battuta del mio professore di lettere, di latino in modo particolare,

l'annuncio che ci saranno altre puntate, o almeno che si propongono altre puntate per questo dibattito. Per carità, io penso che quando si solleva un problema è giusto affrontarlo, discuterlo con molta serenità. Credo, però, che sarebbe utile per tutti che questa serenità venisse utilizzata utilizzata approfondendo alcuni elementi. Voi sapete che Rifondazione Comunista, su una vicenda che è stata molto richiamata e che, in qualche modo, viene collegata al cosiddetto caso Visco (mi riferisco alla vicenda UNIPOL), non ha aspettato intercettazioni, né valutazioni della magistratura, né altro. Dicemmo allora che ritenevamo non opportuna, sbagliata una simile operazione. Voglio ricordare però adesso, visto che è stato fatto riferimento anche ai pronunciamenti della magistratura, che nella richiesta di archiviazione l'ipotesi secondo cui il trasferimento degli ufficiali milanesi sarebbe stato richiesto da Visco in relazione alla loro attività di indagine sulla vicenda UNIPOL è definita dal magistrato: «Nulla più che una illazione priva di riscontri». Mi riferisco al testo. Non pretendo di avere la capacità di lettura dei testi giudiziari

debba intendersi come un dato di illegittimità che ha un riferimento politico, non giuridico.

il reato di abuso di ufficio, seppure in forma soltanto tentata. Se così stanno le cose, continuiamo pure a discutere, abbiamo - credo - tutti la consapevolezza che vi sono stati atti politici compiuti dal vice ministro Visco nell'astenersi, anzi nel restituire la delega alla Guardia di finanza. quanto ho visto anche dagli ordini del giorno, penso che in quest'Aula ciascuno sia libero di giudicare le opinioni espresse da chiunque e anche di criticarle; però, davvero sconveniente che quest'Aula venisse chiamata ad esprimere una censura nei confronti delle opinioni che anche un Vice ministro può esprimere in qualsiasi circostanza, purché non lesive della dignità di altre persone e non offensive della sovranità della legge e della legittimità costituzionale. stanti così le cose, dobbiamo prendere atto di ciò che la magistratura ha detto, assumendo un atteggiamento di grande rispetto nei confronti di quello che la magistratura amministrativa dovrà dire un riconoscimento profondo a quanto il Ministro dell'economia e delle finanze ci ha detto e a quanto il Governo ha rivendicato in termini di autonomia e di legittimità della decisione politica di sostituire il comandante della Guardia di finanza. Tra l'altro, colgo l'occasione buon lavoro al nuovo comandante generale D'Arrigo e a tutta la Guardia di finanza, che sta dimostrando, in continuità con il suo operato e con la sua storia, un'azione importante in direzione del recupero di ingenti somme dall'evasione fiscale.

compattamente e convintamente voterà contro le mozioni e gli ordini del giorno presentati.

con abilità, ha eluso il problema parlando della politica fiscale del Governo. Oggi parliamo d'altro, signor Ministro: la sconcertante vicenda Visco‑Speciale, culminata, il 1° giugno scorso, nell'illegittima rimozione, decisa dal Governo, del comandante generale della Guardia di finanza, generale Speciale, ritorna in quest'Aula, dopo l'ormai famosa seduta del 6 giugno, durante la quale il ministro Padoa-Schioppa, nella sua relazione, si scagliò contro il generale, utilizzando argomenti, aggettivi e accuse ai più apparsi offensivi, nei confronti sia del generale sia dell'intero Corpo della Guardia di finanza. Non è vero, signor ministro Chiti, che da allora non è accaduto niente di nuovo: dal 1° giugno ad oggi vi sono stati almeno tre passaggi che possiamo considerare nuovi. Il primo: il generale Speciale, dopo aver rinunciato alla nomina della Corte dei conti, ha presentato una querela contro il ministro Padoa-Schioppa per diffamazione pluriaggravata. Il secondo: la procura della Repubblica di Roma ha iscritto l'onorevole Visco nel registro degli indagati per i reati di abuso d'ufficio e minacce nei confronti del generale Speciale ed ha concluso l'istruttoria, richiedendo al GIP l'archiviazione del procedimento, definendo, però, l'agire di Visco di Visco illegittimo. Il terzo: pende ancora davanti al TAR il ricorso di Speciale, che ha chiesto il suo reintegro; su questa decisione potrebbe pesare il contenuto del nulla osta alla sua sostituzione rilasciata dalla Corte dei conti. Secondo quanto pubblicato su un giornale certamente non vicino ad Alleanza Nazionale, ossia «la Repubblica», la Corte dei conti ha dato il nulla osta per ragioni d'urgenza, chiarendo che il decreto di nomina dell'attuale comandante, generale D'Arrigo, non poteva dare per implicita la sostituzione di Speciale, perché questo non è ammissibile ed è contro quanto prescrive la Costituzione all'articolo 97. Non ci permettiamo - non l'abbiamo mai fatto - di commentare le conclusioni cui è giunta la procura di Roma, ma nella motivazione della richiesta non possiamo non cogliere quella che ci è sempre apparsa sin dall'inizio come la vera sostanza politica che ci riguarda e su cui il Senato è chiamato a pronunziarsi. Cosa hanno sostenuto, in estrema sintesi, i La condotta del Vice ministro è illegittima, ma non illecita. L'onorevole Visco ha posto in essere una condotta adatta ad ottenere trasferimenti di alcuni ufficiali della Guardia di finanza, ma i magistrati romani hanno accertato che il Vice ministro non aveva alcun potere: il potere decisionale in materia di impiego è attribuito al comandante generale. Restano oscuri i motivi che hanno spinto Visco ad esercitare indebita pressione su Speciale per ottenere trasferimenti di ufficiali che avevano ricevuto, così come il generale Speciale, ripetuti encomi da parte di Visco stesso e della magistratura milanese. Dall'encomio siamo passati all'accusa di golpisti

bensì in un consesso politico e quanto è detto basta e avanza per chiedere al Governo di cacciare Visco da Vice ministro. In sostanza, i fatti nuovi riconfermano l'inopportunità politica che il Vice ministro rimanga al suo posto. Riteniamo insufficiente il fatto che gli siano state congelate le deleghe sulla Guardia di finanza: un Vice ministro che si è macchiato di azioni e comportamenti illegittimi non può restare al suo posto: deve dimettersi e, se non ne ravvisa da solo la necessità, deve essere allontanato. A tale proposito, ci sorprende l'atteggiamento di un autorevole rappresentante del Governo, nonché segretario nazionale di un partito, l'onorevole Di Pietro, che, dopo aver detto che Visco doveva andarsene, ha cambiato idea. Io stimo molto il collega collega Formisano, ma oggi è stato pirandelliano, ha dovuto fare mille parti in commedia per difendere una posizione nella quale non crede nemmeno lui. È venuto alla Conferenza dei Capigruppo, ha chiesto il dibattito, ha detto che voleva il dibattito perché Visco doveva andare via ed è venuto in Aula a dire che invece era rimasto convinto dalle dichiarazioni del Ministro. Non vorremmo che anche questioni di principio, come quelle legate alla vicenda Visco-Speciale, fossero oggetto di mercanteggiamento tra esponenti di Governo. C'è una necessità di trasparenza e di moralità che prescinde da vicende giudiziarie. Per non far parte di un Governo non è necessario che ci sia una condanna penale: basta quanto appurato dai magistrati. Visco ha tenuto comportamenti mendaci nei confronti degli inquirenti e comportamenti illegittimi nei confronti del generale Speciale, aggravati dal fatto che erano giustificati dal voler tutelare l'interesse della propria parte politica a scapito dell'interesse generale della Nazione. Ha persino mentito nel corso dell'interrogatorio dei pubblici ministeri, raccontando circostanze palesemente false. Al Gruppo di Alleanza Nazionale importa solo l'aspetto squisitamente politico; la magistratura farà - come giusto - il resto. Visco, però, deve lasciare il Governo. Il Governo ha caricato il dibattito di oggi - importante, non c'è dubbio oltre ogni logica, lasciando intendere alla propria maggioranza che se passa la mozione dell'opposizione cade il Governo. Non è così. Tanti sono i motivi perché Prodi cada, e faremo di tutto perché ciò accada. Ma un Vice ministro può essere sostituito: è già accaduto ed accadrà ancora. Se invece sono i DS che con il loro *leader* ravvedono la necessità che Visco debba restare al suo posto perché diversamente cadrebbe il Governo, se questa maggioranza è così debole ed il Governo è altrettanto debole

il ministro Padoa-Schioppa, dando il via alla sessione di bilancio, ha detto tante cose inaccettabili, una in particolare: la scorsa legislatura si è conclusa con l'incoraggiamento all'evasione fiscale. L'affermazione si commenta da sola, ma vogliamo tornare all'ordine del giorno di questa sera. Il Ministro ha difeso fortemente il suo Vice, il che sarebbe legittimo, anzi è anche sotto certi aspetti apprezzabile, ma lo ha fatto in un modo così strano, così forte, così fuori da ogni logica, da apparire non la difesa di un collaboratore, bensì quella di un complice: si ha l'impressione di avere di fronte dei complici che si danno la mano l'uno con l'altro. Tra poco la maggioranza voterà contro le mozioni presentate dal centro-destra, ma non ha avuto il coraggio di presentare una mozione di sostegno.

potevate dire: udita la relazione del ministro Chiti, la approviamo. Non ci sono precedenti in materia, è il primo caso che una maggioranza si presenta ad un dibattito politico di tale importanza senza presentare un proprio documento. È di una gravità inaudita, che non dovrebbe trarre in inganno, non dico la pubblica opinione e nemmeno noi dell'opposizione, ma chi siede sui banchi del Governo. Non state difendendo il vostro Governo nemmeno con un documento, perché siete anche voi - mi si passi il termine certamente non parlamentare - schifati degli atteggiamenti di questo Governo. PASTORE *(FI)*. Bravo! MATTEOLI *(AN)*. Allora, vogliamo rivolgere un appello alla coerenza a coloro che hanno condiviso con noi l'opportunità del dibattito e in un primo momento anche il contenuto delle mozioni: non lasciatevi intimorire dai ricatti, non lasciate trionfare l'ipocrisia, votate a favore delle mozioni del centro-destra, ne va della vostra dignità di parlamentari.

Presidente, con tutto il rispetto nei confronti del ministro Chiti, ci saremmo attesi la presenza del ministro Padoa-Schioppa, anche perché riteniamo questa seduta il secondo tempo di una partita che non si è ancora conclusa. Ricordiamo ancora le parole del Ministro, che ha accusato in quest'Aula il generale Speciale di aver quasi gestito la Guardia di finanza come un Corpo autonomo, di non avere avuto rispetto nei confronti della politica e del Governo, di avere esagerato nelle attribuzioni, nelle promozioni e nei trasferimenti gestendo la Guardia di finanza come se fosse una cosa propria.

I magistrati - non il Gruppo Forza Italia - hanno accertato che «la condotta di Visco appare illegittima e questo ufficio ritiene che il Vice ministro abbia posto in essere una condotta in violazione di specifiche norme di legge. Il quadro normativo che disciplina il trasferimento degli ufficiali della Guardia di finanza è estremamente chiaro, in materia il Vice ministro non ha alcun potere». Quindi, la dimostrazione *per tabulas* attraverso un'indagine correttamente compiuta dalla procura di Roma che il vice ministro Visco aveva abusato del proprio ruolo, avendo esercitato indebite pressioni nei confronti del comandante della Guardia di finanza. Ci saremmo attesi la presenza del Ministro per ascoltare la replica la replica di un uomo che non ha lesinato parole pesantissime nei confronti di un comandante generale invece elogiato qualche giorno prima dallo stesso vice ministro Visco, quando il 4 aprile, alle 13,48, un'agenzia affermava che, secondo le parole d'apprezzamento del vice ministro Visco, si ringraziava il generale Speciale per l'impegno e il non aver abbassato la guardia nel contrasto all'evasione. Da un lato, quindi, si rimuove il generale Speciale perché si sostiene che non ha assolto compiutamente il proprio ruolo, dall'altro lato, mentre qualche giorno prima lo si elogiava, lo si rimuove chiedendone lo spostamento alla Corte dei conti. Avremmo voluto ricordare al ministro Padoa-Schioppa come diverso sia stato il comportamento di alcuni ex Ministri del centro-destra, i quali, soltanto per essersi resi protagonisti di alcune espressioni, anche disdicevoli, non opportune, ma soltanto riconducibili al linguaggio politico dell'espressione del pensiero, soltanto in forza di quegli atteggiamenti, con grande senso di responsabilità e per non arrecare una frattura tra il corpo elettorale e le istituzioni, che invece voi avete determinato con la rimozione di Petroni e del generale Speciale, hanno avuto il coraggio di dimettersi. Signor Presidente, colleghi della maggioranza, ci si dimette quando, ricoprendo ruoli istituzionali, ci si rende conto che con il proprio comportamento si lede il prestigio e l'autonomia delle istituzioni, e i nostri ex Ministri lo hanno fatto.

in forza della quale si attesta che indubbiamente si è trattato di un'interferenza indebita nell'ambito delle prerogative che la legge attribuisce al comandante generale, dinanzi all'accertamento giudiziario, esaustivo, che il vice ministro Visco ha compiuto un'interferenza e ha abusato del proprio ruolo, ha quindi compiuto un atto illecito, utilizzando il ruolo istituzionale che

stupore del Governo per la richiesta di questo dibattito perché «nulla è cambiato». No! È cambiato qualcosa. È cambiata la verità, acclarata dai magistrati della procura di Roma, che ha confermato come le nostre lagnanze fossero veritiere, fondate. È cambiata la verità.

Oggi, quella coalizione elettorale, quell'opposizione di una volta, unita soltanto per battere qualcuno, ripercorre quello scenario, perché in assenza di una capacità di governo del Paese non ha nemmeno la forza e il coraggio di presentare un proprio documento sul quale trovarsi unita. È la prima volta che succede in questa legislatura e non era mai accaduto nella nostra. Non presentate un documento perché avete paura di non avere i numeri per approvare la relazione del ministro Chiti. Ecco la vostra crisi. Non avete questo coraggio perché avete paura di sfiduciare il ministro Chiti, come avete sfiduciato il ministro Parisi sulla politica estera. Mi accingo a concludere, signor Presidente. La difesa del vice ministro Visco appartiene alla difesa disperata di un Governo che si arrocca ad applaudire dissennatamente le dichiarazioni del Ministro dell'economia che elogia una finanziaria che i cittadini non vogliono e del cui rifiuto il Governo non si sta accorgendo di quanta delusione vivano quotidianamente per la politica economica di un Governo che, anziché eliminare gli sprechi e ridurre la spesa pubblica, utilizza le maggiori entrate fiscali soltanto per "allattare" il partito della spesa pubblica che noi invece intendiamo contrastare.

Il senatore D'Onofrio, nell'illustrare la sua mozione, ha parlato di tre profili: un profilo giuridico-penale, uno giuridico‑amministrativo ed uno politico.

e, nell'affrontarlo, utilizza elementi che sono parte della motivazione che è stata posta alla base della richiesta di archiviazione della procura di Roma

quello che ha scritto la procura di Roma: «l'ipotesi secondo cui il trasferimento degli ufficiali milanesi della Guardia di finanza sarebbe stato richiesto dall'onorevole Visco in relazione alla loro attività d'indagine sulla vicenda UNIPOL» è definita dalla procura della Repubblica «nulla più che una illazione priva di riscontri».

richiesta di archiviazione della procura di Roma. Allora, anche su questo punto voglio ricordare a lei e a tutti i colleghi che la procura osserva che non c'è alcun rilievo penale, in quanto gli atti compiuti dall'onorevole Visco non si configurano come abuso d'ufficio, poiché non vi sarebbe prova di dolo intenzionale.

Certo - non ho difficoltà a riconoscerlo - è anche il risultato di alcune misure importanti che sono state adottate nell'ultima finanziaria

di aver condotto con testardaggine un'azione importante nei confronti dell'evasione fiscale e di aver ascoltato anche i suggerimenti e le proposte che abbiamo avanzato, per far sì che la lotta all'evasione fiscale contenesse elementi di prevenzione, colpisse e snidasse le grandi evasioni e fosse accompagnata anche da un rapporto costruttivo con i contribuenti. Non a caso ci siamo ci siamo battuti per riaffermare i diritti dello Statuto del contribuente. Questa finanziaria è la prima nel nostro Paese a non contenere nessuna norma retroattiva, nessuna di

voi non potete assolutamente evadere questo discorso. Non potete parlare solamente di Visco e non parlare, invece, di un

ha avuto la responsabilità istituzionale di rassegnare le deleghe e prendendo atto di quanto ha riferito il ministro Chiti, noi poniamo con forza al Governo la (congelamento o meno delle deleghe) deve risolvere un problema. Noi avvertiamo la necessità che nel decreto-legge e nella legge finanziaria

venga recuperata. Siamo convinti di dover offrire una prova importante di fiducia verso questi servitori dello Stato, che combattono la battaglia per rendere il nostro fisco più equo.

ha stabilito di mettere in votazione queste mozioni in ordine cronologico e l'Assemblea ha convenuto. Questa mattina il presidente Angius, con la condivisione di diversi colleghi di maggioranza e opposizione, ha posto alla Presidenza la questione

avverto gli onorevoli colleghi che, conformemente alla prassi del Senato, l'esito di ciascuna votazione non sarà ostativo alla votazione degli strumenti successivi, che si intenderanno messi ai voti per le parti palesemente non precluse né assorbite.

La seduta è ripresa. Colleghi, raccomando proprio la compostezza, perché, anche in un dibattito così teso come è stato quello di oggi, debbo dire che il comportamento

che ha offeso un intero popolo, che è asse portante dell'economia e della democrazia di questo Paese.

vice ministro Visco ha reso in una manifestazione pubblica, a proposito della cultura media dei cittadini della Regione, che a suo dire sarebbero caratterizzate da una pregiudiziale ostilità allo Stato.

io credo che chi ha governato fino ad un anno e mezzo fa questo Paese, e quindi anche quel territorio che chiamiamo Veneto, forse avrebbe dovuto rispondere di più alle attese degli elettori del Veneto portando a casa più risultati, per esempio sul piano del federalismo fiscale, di quelli che abbiamo visto sul territorio. Noi crediamo di far parte di un Governo che su questi temi si sta impegnando. *(Vivaci

insieme con il vice governatore Zaia, sono esponenti di Forza Italia e della Lega Nord, chiedono maggiore autonomia per la Regione attraverso l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 116 della Costituzione che è quello che la vostra riforma abrogava. Quindi avete preso in giro i cittadini veneti. del vice ministro Visco, che io non chiedo, da parlamentare del Veneto, che sia censurata una sua affermazione da sociologo.

succede che tanti di destra, di centro e di sinistra, signor Presidente. Vorrei ricordare alla senatrice Valpiana che lo Statuto della regione Veneto parla

orgogliosi di essere italiani nella misura in cui ciascuno di noi è orgoglioso delle proprie radici. Quindi, da toscano, insieme a tutti i toscani di quest'Aula,

dopo l'intervento del collega Palma, la sintesi dell'accaduto della seduta di questa mattina in occasione del voto sulla mozione Malpensa.

un voto articolato capoverso per capoverso, nella parte dispositiva e nella parte anche motiva. Poi la Presidenza aveva suggerito che la parte motiva si votasse nella sua interezza e si era accettato questo suggerimento, ma tutto rimaneva immutato in proposito all'intesa dell'Aula sulle modalità di voto, capoverso per capoverso, del dispositivo.

dispositiva nella sua interezza, ha erroneamente registrato il voto favorevole di Forza Italia. Infatti, in quel momento il mio Gruppo riteneva si stesse votando soltanto il primo capoverso della mozione, e non altro.

si votano prima le mozioni più distanti rispetto alle altre, in maniera da evitare che vi siano assorbimenti e scostamenti. Comunemente, all'unanimità, l'Assemblea ha stabilito

perché, in una delle tante circostanze, è accaduto che abbiamo espresso un voto senza sapere che cosa stessimo votando. Non le ricordo la circostanza, così evitiamo polemiche.

Come ricorderà, abbiamo votato per parti separate, per cui, alla fine, sono risultati approvati un comma della premessa ed il terzo comma del dispositivo.

sull'Alitalia? La Presidenza ha letto un annunzio, che è uguale a quello dato questa sera. Mi consenta di leggerlo, tanto sono due righe: «L'esito di ciascuna votazione non sarà ostativo alla votazione degli strumenti successivi, che si intenderanno messi ai voti» (quindi, non si tratta di approvati o non approvati, ma messi ai voti, fase ancora «per le parti palesemente non precluse né assorbite». È evidente che il "palesemente" è un giudizio discrezionale del Presidente, ma non è questa la mia osservazione. La mia osservazione è nel metterlo ai voti, io che voto non so effettivamente lei che cosa abbia considerato assorbito o precluso, quindi di fatto voto senza saperlo. Io senatore voto senza sapere che cosa il Presidente domani deciderà essere precluso o assorbito. Questo, signor Presidente, non può accadere. Lei, ripristinato questa prassi, che è antecedente a quella della sospensione e della decisione. Non dico che non mi vada bene: anche questa è una soluzione che ci consente di proseguire. Però, signor Presidente,

Però questa mattina il presidente Angius ha introdotto, seppure con molto garbo e a titolo personale, tale questione, dicendo che non possiamo andare avanti così, perché votare in questo modo alla fine stravolge il senso complessivo della proposta che fa un senatore con le parti separate, quelle assorbite e quelle precluse: è una cosa che non funziona.

una riflessione nella Conferenza dei Capigruppo o nella Giunta per il Regolamento perché oggettivamente così avanti non possiamo andare. Ora, Presidente, se se lei mi usasse la cortesia di leggere la mozione che abbiamo approvato e poi gli ordini del giorno di questa sera, troverebbe che oggettivamente ci sono delle parti che possono essere palesemente o non palesemente ritenute assorbite o precluse. Allora, ancora una volta questa sera abbiamo votato e fortunatamente abbiamo respinto tutto, quindi il problema in sé non c'era, però la questione esiste.

quando abbiamo finito di votare si sappia esattamente il Senato che cosa ha approvato. Non volevo dire nulla di più, signor Presidente, in maniera costruttiva. L'ho detto adesso, a fine seduta, e la ringrazio, ma secondo me

*(Misto-LD)*. L'invito è respinto, perché non vorrei che qui passasse una tesi sbagliata. Io ho molto rispetto per le capacità causidiche del senatore Boccia, ma le cose non stanno come racconta lui.

i lavori preparatori della Giunta per il Regolamento relativamente alla possibilità, prevista dal Regolamento, di votare per parti separate. Che cosa dice il nostro Regolamento? Afferma che è un diritto; un diritto che è stato espressamente voluto dal legislatore quando ha regolamentato i nostri lavori

In un solo caso ciò può avvenire: quando l'Aula respinga la richiesta di votare per parti separate. Non vorrei che adesso si introducesse un argomento surrettizio, fasullo e che non c'entra niente con quello che è successo qui dentro. Dobbiamo stare attenti a rispettare il nostro Regolamento perché è la garanzia per tutti.

frequentatore del Parlamento e sa benissimo che il problema, quando si presentava, veniva risolto dalla coesione che le maggioranze avevano al proprio interno.

spero proprio che ella voglia fare riferimento al fatto che il Regolamento non è che possa essere cambiato per contingenze momentanee, ma deve essere variato al momento in cui una difficoltà si presenta con costanza.

dall'enorme diversità della maggioranza rispetto alle decisioni da prendere sia in politica estera che in politica interna che in politica economica, e chi più ne ha più ne metta. Non vorrei che questo portasse come conseguenza, rispetto alle attese e alle proposte del senatore Boccia, una modifica del Regolamento. In questo caso, infatti, cosa si dovrebbe fare? Parlare di modifiche del Regolamento

non è qualcosa che viene accettato. Il senatore Boccia all'inizio del suo intervento, credo per cattivo uso dell'italiano, ha detto: «noi abbiamo accettato». Il Regolamento non si accetta,

nel senso che la discrezionalità del Presidente nel momento in cui si pone il problema in Aula del voto per parti separate riguarda solo il suo giudizio se si riferisca a più soggetti od oggetti, o sia comunque suscettibile di essere distinto, in quel caso il Presidente può dire che non ci sono le condizioni, ma il rifiuto non è previsto.